Colleghi, se vogliamo dare ordine ai nostri lavori, che sono complessi e numerosi, e terminare, come entrando ognuno chiede, sarà bene cercare di prestare un minimo di attenzione. Comunico che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è autorizzata a convocarsi oggi, alle ore 14,15, per questioni attinenti alle materie di sua competenza.

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale in senso ampio. Il provvedimento contiene misure tese a rafforzare i risultati

n. 90 del 2008 aveva introdotto un modello per la gestione dell'emergenza dei rifiuti in Campania incentrato sulla nomina di un sottosegretario di Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuato nella persona del dottor Guido Bertolaso.

legislativo che tenga conto di queste esperienze e disegni per il futuro un modello normativo che possa essere eventualmente - ci auguriamo mai auguriamo mai - utilizzato in caso di insorgenza di situazioni di crisi analoghe, in modo da non dover operare ogni volta con una decretazione specifica regione per regione o territorio per territorio,

per garantire l'osservanza della normativa in materia di rifiuti con i relativi strumenti sanzionatori, compreso il commissariamento dei Comuni e delle Province inadempienti, relativamente alle norme di competenza dei singoli enti. esame sono altresì inseriti norme finalizzate a velocizzare la rimozione dei rifiuti ingombranti, interventi per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e la previsione della corresponsione di emolumenti al personale militare impiegato,

una significativa quantità di ore di straordinario che devono essere remunerate. Quindi, anche in questo caso questo tipo di problema emerso trova risposta nel provvedimento oggi all'esame di questa Per tutti i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti il decreto-legge inasprisce poi le sanzioni attualmente previste per alcune violazioni della normativa in materia di rifiuti. È prevista una campagna informativa per il corretto comportamento in materia di smaltimento di rifiuti e per la conoscenza delle nuove sanzioni introdotte, cittadini, anche dal punto di vista economico, la convenienza del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata nonché ad introdurre l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo. Infine, sono introdotte modifiche alle norme che consentono l'incentivazione dell'energia prodotta dai termovalorizzatori, al fine di facilitare l'equilibrio dei piani finanziari necessari alla loro realizzazione, con particolare attenzione a quegli impianti connessi a situazioni di emergenza già dichiarata prima della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, Passando all'analisi del provvedimento in maniera più approfondita, troviamo all'articolo 1 misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti da imballaggio. L'articolo autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, una serie di attività. Nello specifico: la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati, allo scopo autorizzati. A questi soggetti viene riconosciuto un indennizzo forfetario a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti,

occasionale e saltuaria di tanti soggetti di piccole dimensioni. Questi ultimi, avendone una remunerazione e un'autorizzazione provvisoria, possono aiutare il sistema ufficiale nella raccolta di grossi quantitativi di imballaggio che si sono prodotti e anche nella raccolta di quell'imballaggio che viene prodotto al momento ma che, se non trovasse questa polverizzata e distribuita capacità aggiuntiva, saltuaria o occasionale, presente sul territorio, andrebbe a intasare intasare i normali flussi di smaltimento che si stanno definendo e costruendo in questa fase commissariale. Un'altra autorizzazione che viene definita, sempre relativamente a questo tipo di nuova attività saltuaria o occasionale, è quella della esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce tali rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati alla allo schema costruito in questi mesi dalla gestione commissariale, vengono anche facilitati con la esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di 2 milioni di euro, sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale competente a valere sul fondo per l'emergenza dei rifiuti Campania. L'articolo 2 L'articolo 2 tratta della rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi e di impianti di gestione dei rifiuti. Questo articolo, per fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti in siti non autorizzati, attribuisce ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti, nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisori e di smaltimento. Per la durata dello stato di emergenza, quindi, i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei titoli abilitativi per i quali è consentito l'affidamento diretto, purché essi siano in possesso della necessaria idoneità tecnica. Detti soggetti sono autorizzati a derogare dalla procedura vigente in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché in materia di bonifica di siti contaminati. Infatti, i soggetti pubblici competenti, informando le autorità sanitarie competenti, individuano - anche in deroga alla normativa vigente - siti di stoccaggio provvisori dei rifiuti, che saranno poi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento. È evidente la *ratio* di questo provvedimento: se dobbiamo uscire (come stiamo uscendo, ormai in maniera evidente) da una situazione di emergenza, abbiamo bisogno di siti provvisori di stoccaggio, in attesa di avere a disposizione gli impianti che tratteranno in via definitiva questa

stesso articolo autorizza il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli stessi. stessi. Anche questo tema è stato abbondantemente evidenziato nelle discussioni nelle Aule parlamentari, in quanto uno dei punti critici, una delle zone opache della gestione dei rifiuti è proprio la loro tracciabilità e il rischio che, all'interno dei flussi

del rapporto di fiducia da ricostruire con i cittadini. Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione di questi siti di stoccaggio provvisorio entro 15 giorni dalla richiesta,

se le autorità che hanno la responsabilità di realizzare questi siti non hanno risposte in tempi certi, subentra il principio dei poteri sostitutivi, che in questo decreto sono assegnati al Ministero dell'ambiente, entro 15 giorni. Il comma 4, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza, autorizza il Sottosegretario di Stato a disporre la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia nonché, sentiti gli enti locali competenti, ad individuare un sito idoneo nel territorio della Regione stessa. Tale nuovo impianto consentirebbe l'eliminazione di oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti, ex CDR, stoccate in numerose aree disseminate nel territorio campano. È di tutta evidenza ai colleghi che l'enorme quantità di materiale combustibile derivato dai rifiuti, stoccato in vario modo, in tante parti della Regione, se non avrà un impianto dedicato, non potrà di certo essere smaltita dagli impianti che sono calibrati e dimensionati per la produzione ordinaria

a individuare il sito, sentiti gli enti locali, e a passare alle fasi di progettazione, costruzione e gestione di questo impianto finalizzato. L'articolo 2-*bis*, concernente l'estensione dell'area di interesse strategico nazionale ad uffici e a sede degli impianti, fa riferimento all'individuazione di aree di interesse strategico nazionale, principio già previsto nel decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, e aggrega a questa definizione anche le sedi degli uffici funzionali alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti. L'articolo 2-*ter*

si intendono autorizzati, per un triennio, lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie di rifiuti urbani presso qualsiasi area di deposito temporaneo, nelle more del funzionamento degli impianti in cui verranno trattati. Il comma 2 stabilisce che l'attuazione della norma interpretata è sottoposta all'autorizzazione comunitaria per una corretta e piena legittimazione. il commissariamento degli enti locali; ne facevamo cenno nelle poche parole introduttive. L'articolo dispone la rimozione, con decreto del Ministero dell'interno (su proposta motivata del Sottosegretario), del sindaco, del presidente della Provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte, sia dei Comuni che delle Province, nel caso di grave inosservanza della normativa in materia di gestione dei rifiuti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Evidentemente - come dicevo in stiamo parlando di gravi inadempienze per le responsabilità e per le competenze di ognuno dei due singoli enti che potrebbero essere oggetto di commissariamento. L'articolo 4 riguarda l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella Provincia di Caserta. Per tutto il periodo dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali, che - come i colleghi sanno - sono previste dalla legge regionale, i Comuni della Provincia di Caserta, che si avvalgono del consorzio per la raccolta dei rifiuti, avviano, anche in forma associata, le procedure per affidare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi di deroghe già previste, con particolari indicazioni in merito all'assegnazione del personale. Vi è un problema di personale che era in carico ai preesistenti consorzi e che deve essere opportunamente distribuito. All'articolo 5 tratta del lavoro straordinario del personale militare. Tale articolo autorizza la corresponsione al personale militare operante presso le strutture commissariali di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, per una spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. L'articolo 6 riguarda la disciplina sanzionatoria, si è svolto un ampio dibattito nel Paese e anche in Commissione. Tale articolo introduce un più rigoroso sistema sanzionatorio per una serie di condotte già vietate dal 152 (codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da contravvenzionali a delittuose (la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose). È un significativo inasprimento delle pene. Come è evidente, l'obiettivo di questa norma è di accentuare la capacità di potere deterrente da parte della disciplina sanzionatoria.

regionale e locale ma di coordinamento complessivo, perché nel momento in cui va in crisi un sistema ne risponde tutto il sistema nazionale. Quindi è opportuno che in questo decreto, sulla base delle esperienze acquisite, si pongano le basi anche per una visione strategica di tipo nazionale. L'articolo 7-*bis*, concernente l'educazione ambientale, di straordinaria importanza dal punto di vista dei dei principi, introduce, in accordo con il Ministero dell'istruzione, l'indicazione di costruire dei programmi di educazione ambientale all'interno delle scuole. L'articolo 8 (Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi) prevede l'assegnazione in comando al Dipartimento della protezione civile di un minimo di 35 unità di personale operativo, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili con l'obiettivo di favorirne la realizzazione in quanto tassello indispensabile per il completamento di un sistema integrato funzionale, in grado di evitare le situazioni di emergenza ovvero di uscire da tale stato. dispone misure urgenti in materia di rifiuti al fine di risolvere le difficoltà riscontrate da operatori nel recupero rifiuti, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare

9-*quater* reca altre misure urgenti in materia di rifiuti. L'articolo 10, in conclusione, è una norma di interpretazione autentica, volta ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nel senso di considerare creditori, quindi pagabili dalla gestione commissariale a scomputo dei crediti delle società affidatarie verso la gestione commissariale stessa, anche le società appartenenti al medesimo gruppo delle società affidatarie che avevano svolto prestazioni come subappaltatori, fornitori o cottimisti per le affidatarie stesse

In particolare, l'articolo 6 desta perplessità in quanto introduce diverse fattispecie di incriminatrici di condotte, peraltro tra loro eterogenee, violative di disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti; tali norme si applicano esclusivamente ai territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, Il problema giuridico, di natura costituzionale, sorge nel momento in cui l'unico territorio interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti è quello della Regione Campania. Tale delimitazione *ratione loci* della sfera di applicazione di norme incriminatrici appare difficilmente compatibile con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce rilevanza penale a una medesima condotta, non già in ragione della sua intrinseca offensività rispetto al bene giuridico protetto, ma unicamente in ragione del *locus commissi delicti*. Quanto a questo profilo di illegittimità, oltre a determinare un'incompatibilità delle nuove nonne con il principio di uguaglianza, esso confligge con il principio di territorialità del diritto penale, diritto penale, sancito dall'articolo 3 del codice penale, che è ritenuto uno dei principi fondativi del sistema penale, diretta espressione del principio della sovranità statuale, sancito dall'articolo 1 della Carta costituzionale. Non si comprende, ad esempio, per quale motivo dovrebbe configurare un delitto abbandonare una lavatrice o un frigorifero in Campania e non nelle acque del Tevere o nei canali di Venezia. La stessa subordinazione dell'applicabilità della fattispecie alla previa declaratoria dello stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992, si ritiene configgere con i principi di tassatività, determinatezza,

ad un mero provvedimento amministrativo la determinazione del contenuto e della sfera di applicazione del precetto. A questo proposito sono intervenute plurime sentenze della Corte costituzionale, la quale ha in più occasioni ravvisato ipotesi di violazione del principio di legalità laddove non sia una legge dello Stato ad indicare con sufficiente precisione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti amministrativi ai quali consegua una sanzione penale (si ricordano, in particolare, le sentenze n. 58 del 1975 e n. 199 del 1993). In particolare, la Consulta ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ogni qualvolta l'amministrazione conservi il potere di modificare o di revocare l'atto al quale sono connessi gli effetti penali, in quanto tale tecnica nomotetica induce incertezza in ordine alla definizione della condotta illecita e sottende un rinvio da parte della legge a un potere subordinato, incompatibile con la riserva di legge in materia penale (la sentenza cui si fa riferimento è la n. 282 del 1990). Un'ulteriore violazione dei principi di offensività, ragionevolezza ed uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma secondo, del resto dalla stessa correlazione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge, tra rilevanza penale della condotta e luogo di realizzazione del fatto, subordinandosi la punibilità alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 l'emergenza ambientale non abbia connotati equivalenti in ogni comprensorio della Campania ed è parimenti evidente come la declaratoria ai sensi della legge del 1992 non possa distinguere area per area, trattandosi di una deliberazione governativa orientata secondo valutazioni generali circa l'andamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Può, quindi, verificarsi che siano gravemente puniti comportamenti posti in essere in luoghi, di fatto, non insalubri o non esposti a rischi ambientali, ma formalmente ricompresi nell'area soggetta alla declaratoria di emergenza, con conseguenti comportamenti criminogeni da parte dei cittadini ed evidente violazione dei principi di offensività, ragionevolezza ed uguaglianza già ricordati. Analoghi dubbi di compatibilità con i princìpi ricordati suscita l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, ove il peculiare disvalore della condotta si radica sulla qualifica soggettiva dell'autore, titolare di un'impresa o responsabile di un ente, con le conseguenze che ne potrebbero derivare in ordine alla quantità di rifiuti che potrebbero essere illecitamente trattati o smaltiti. L'assenza di qualsiasi richiamo, nella norma suddetta, a quello che deve essere considerato un requisito modale indefettibile della condotta, ossia l'aver agito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o dell'ente, rischia di violare i principi di ragionevolezza, eguaglianza e personalità della responsabilità penale (articoli 3 e 27, comma secondo, della Costituzione), configurando così una forma di colpa

volete che sia sospesa la seduta per dieci minuti per riflettere, per trovare l'equilibrio e la tranquillità o lasciamo parlare la senatrice Della Monica?

dall'articolo 3, che prevede la rimozione del sindaco, del presidente della Provincia e di una serie di organi rappresentativi delle autonomie locali. va ad inserirsi in un sistema già strutturato, contemplato dagli articoli 141, 142 e 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nel corso della discussione che è stata svolta alla Camera, sono state avanzate varie perplessità rispetto all'articolo 3, soprattutto riguardo all'*iter* del commissariamento e dello scioglimento degli organi, poiché la formulazione originaria della norma era assai generica e poteva, sotto questo profilo, destare perplessità e risultare pericolosa. La nuova formulazione, anche a seguito di interventi costruttivi del Partito Democratico, appare sicuramente migliorativa, perché prevede un percorso graduale. Ciò nonostante ritengo che ci siano due profili che esprimono gravi limiti: il primo è la disarmonia con cui la norma si inserisce nel sistema generale della rimozione degli organi degli enti locali il secondo è l'ancoraggio oltre che a violazioni di legge, peraltro non necessariamente previste come gravi e reiterate, anche a violazioni di ordinanze della Protezione civile, che sono problematiche dal punto di vista costituzionale e che possono comportare gravi possibilità di violazione del principio di legalità. Rimane inoltre, a mio avviso, ulteriormente problematica la questione della rimozione con un *iter* sommario dei componenti dei consigli, ossia di soggetti che sono eletti da corpo elettorale. Non si può confondere in ogni caso, quindi, l'efficacia del provvedimento di rimozione con un principio democratico che è alla base di questi organismi. Passando poi all'articolo 6, è innanzitutto censurabile dal punto di vista politico che si finisca per affrontare il problema e il tema delle sanzioni ambientali con provvedimenti manifesto che sono avulsi da un sistema Il senatore Casson ha espresso forti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, che condivido; vorrei mettere in rilievo che l'inefficacia costituzionale delle norme che si vogliono introdurre finisce col determinare un aggravio inutile del sistema investigativo e giudiziario: lascia più perplessi perché non si comprende per quale motivo, malgrado l'*iter* che si è svolto alla Camera, non si voglia estendere il medesimo sistema sanzionatorio su tutto il territorio nazionale. La conseguenza di questa normativa è che, mentre per tutto il territorio nazionale i medesimi comportamenti sono sanzionati dall'articolo 255 della legge sull'ambiente, e quindi sono puniti esclusivamente con una sanzione di carattere amministrativo, in Campania costituiscono delitto e oltretutto con una assimilazione dello scarico di rifiuti ingombranti allo scarico dei rifiuti tossici. L'irragionevolezza di queste normative comporterà necessariamente il ricorso alla Corte costituzionale, che può essere richiamata anche sotto un altro profilo. non necessariamente tutti i cittadini devono conoscere le ordinanze vigenti su un determinato territorio che costituiscono poi la base perché si possa applicare un diritto penale speciale.

Per questi motivi chiedo nuovamente che il Governo possa prendere in considerazione l'ipotesi non di abolire la norma, cioè il delitto,

una normativa molto semplice, cioè quella che attribuiva alla competenza delle procure distrettuali la possibilità di intervenire su questo tipo di reati. In questo modo temo che si vogliano creare creare dei *vulnus* costituzionali in maniera da favorire una sorta di federalismo, anche penale e processuale penale, che sicuramente contrasta

testimonia la crisi, la difficoltà che attraversa questo Paese nell'affrontare una materia di grande delicatezza.

di questo Paese sono sotterrati all'interno del territorio della Campania. Vorrei cogliere l'occasione odierna per sottolineare che non possiamo andare avanti con continui decreti.

propria legge, che fa riferimento alla provincializzazione. Nonostante ciò, il Governo Berlusconi e il sottosegretario Bertolaso, oltre a individuare discariche

sull'utilizzo delle cave abbandonate nella Regione Campania. A tale questione non si mette mano, ma si preferisce essere presenti continuamente a Napoli perché probabilmente lì ci sono difficoltà

tragica. È vero che sulla materia ambientale c'è un ritardo sul piano più generale, ma c'è anche un senso di responsabilità che, come Parlamento, dobbiamo recuperare. Basti ricordare che nelle numerose audizioni della Commissione ambiente, presieduta dal senatore D'Alia, abbiamo avuto alcune proposte da Federambiente e dalla società d'imprese ANIDA, che

Desidero altresì rassicurare chi ha temuto per la continua presenza di Berlusconi a Napoli anche dal punto di vista culturale. Qualcuno si è preoccupato per la storia e la cultura di Eduardo e qualche altro per la sceneggiata napoletana. A me sembra si possa parlare più di una sceneggiata e di *spot* continui, dove più che rappresentare il senso dello Stato si rappresenta l'impotenza dello Stato in proposito, attraverso proroghe continue un'altra scadenza fino al 2009. Penso che dobbiamo rispondere con una capacità progettuale. Ho ascoltato la relazione del senatore Fluttero

Credo che la logica sia quella dei commissariamenti, dello svuotamento del territorio e delle rappresentanze sul piano della democrazia. Credo che con questo ennesimo decreto e con questo ennesimo ritardo rischiamo moltissimo la credibilità dello Stato, al di là della maggioranza e dell'opposizione. Su tale problema ci vuole la massima solidarietà, la massima capacità di recuperare una

aree. Basterebbe rassicurare i cittadini della Campania, e mi rivolgo alla collega senatrice Armato. Questi, non potendo sversare i rifiuti ingombranti nella regione Campania, Campania, si attrezzano per portare i rifiuti fuori della regione. Lì cosa fanno? Restituiscono i rifiuti del Nord arrivati in Campania! Come si può immaginare un articolo del genere?

una concezione dello Stato come di una proprietà privata. Chiedo anche un senso di responsabilità da parte dei colleghi senatori della Campania. Perché il cittadino della Campania deve essere considerato diverso dal resto del Paese, anche rispetto a fenomeni

di oltre 409 cave, abbandonate e dismesse sul territorio regionale, commissariate dal Governo nazionale, e quindi dal Governo Berlusconi, ovviamente nel corso degli anni passati. Bisogna affrontare questa materia in modo organico e complessivo. Non possiamo più affrontarla in questa maniera, non solo perché non riusciremo a risolvere il problema

questo aspetto con grande determinazione. Tra l'altro, con i colleghi del PD e con altri colleghi dell'opposizione, abbiamo proposto una serie di emendamenti e di ordini del giorno migliorativi se, come vediamo dall'inizio di questa legislatura, è inutile presentare emendamenti. Si chiede un confronto per migliorare i decreti e le leggi, ma poi puntualmente ogni proposta viene respinta. Dobbiamo avere un senso di grande responsabilità

sperperano una grande responsabilità, senza grandi controlli, con deroghe infinite rispetto alla normativa e con l'unico ricavo del disorientamento delle comunità e dei cittadini. Il problema sta tutto lì.

a mio parere si continua a vivere nella medesima condizione. Anche rispetto a questa prospettiva, per un certo verso si è chiesta la collaborazione delle istituzioni territoriali. L'altro ieri, nel corso della conferenza stampa di fine anno, il Presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni delle istituzioni territoriali. Le istituzioni non agiscono a comando e secondo il comodo di chi ha una responsabilità politica o, in questo caso, istituzionale.

avrei svolto partitamente, articolo per articolo, la dimostrazione di tale mancanza di necessità - ma, soprattutto, siamo di fronte ancora una volta al al superamento di norme autorizzative e a deroghe in materia di appalti pubblici e di contratti. Ciò non serve al Paese, né alla Campania: non serve a nulla e a nessuno. Non possiamo immaginare che

il senatore De Luca; vorremmo tornare a previsioni legislative che consentano agli enti locali di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza senza essere senza essere esautorati o falcidiati nei loro poteri; nello stesso tempo, vorremmo una legislazione che consenta anche di prevenire quanto accade. Ancora una volta, invece, il decreto non dà risposte in termini di ordinarietà soprattutto, non dà le risposte che la Campania si aspetta. In particolare, come si svolgerà l'ordinata raccolta dopo l'emergenza? Come saranno gli smaltimenti? La raccolta differenziata avrà sbocchi o non li avrà? Come verranno smaltiti ci dicono che ce ne sono tanti, ma nessuno ne parla mai Le bonifiche dei siti inquinati come avverranno? Di quali controlli effettivi si avvarrà il sistema? Come si eviteranno le infiltrazioni della camorra dentro il sistema?

E sarà solo il ritorno alla vita normale a dirci se avremo gestito bene l'emergenza. Credo che non si possano continuamente inventare decreti, magari con strane norme (come quella contenuta nell'articolo 6, che fa pensare ad una specie di federalismo nel diritto penale)

Presidente, onorevoli senatori, questo provvedimento, tra tutti quelli che hanno riguardato l'emergenza rifiuti in Campania, è quello che oggettivamente lascia maggiormente insoddisfatti. In esso, purtroppo, l'emergenza dei rifiuti in Campania c'entra veramente poco. È un pretesto. È semplicemente la scusa per costruire un decreto *omnibus*, dove inserire di tutto e di più. E poi il metodo: ancora una volta un provvedimento in Aula immodificabile da parte del Senato. Il Presidente della Commissione ambiente ha lamentato pochi giorni fa questo modo di procedere, ma non si può non registrare persino l'inutilità delle sue osservazioni. Di emendamenti e di lavoro parlamentare, in questa conversione, ci sarebbe stato bisogno. Basterebbe guardare i primi due articoli. Da un lato si allargano le maglie del controllo su un territorio che non può assolutamente permettersi cedimenti ulteriori sull'argomento attraverso procedure semplificate nella raccolta e nello smaltimento, dall'altro non si coglie che l'affidamento diretto del trasporto dei rifiuti tornerà ad esporre gravemente gli amministratori locali a pressioni e condizionamenti. Infatti, cos'altro dovrebbe rappresentare l'autorizzazione alla raccolta e allo smaltimento degli imballaggi come occupazione saltuaria o occasionale? Oppure la deroga che consente l'affidamento diretto per la rimozione e il trasporto dei cumuli di rifiuti in apposite aree attrezzate quali siti di stoccaggio provvisorio, anch'esse in deroga alla vigente normativa? Ho come la sensazione che si riallarghino pericolosamente le maglie dei controlli di legalità e che rischiamo di assistere, nuovamente, ad uno scontro tra interessi contrapposti non del tutto legittimi. Così come appare poco convincente un differente trattamento riservato potenzialmente ad aree con problemi simili. Guardate questo decreto-legge: da un lato le prescrizioni sanzionatone si allargano ad ogni territorio in cui vige lo stato di emergenza, dall'altro i cosiddetti «vantaggi» previsti dal provvedimento si circoscrivono e si limitano. La verità è che non c'era bisogno di un decreto-legge per compensare il lavoro straordinario dei militari, dei militari, per svolgere campagne informative o di formazione scolastica senza costi aggiuntivi o per qualche comando che riguarderà alcuni Vigili del fuoco. si fosse voluto metter veramente mano ad un decreto-legge per aiutare pezzi importanti del Paese, si sarebbe dovuto estendere la possibilità della salvaguardia dei livelli occupazionali a tutto il territorio italiano; si sarebbe potuto ricorrere alle risorse della Cassa depositi e prestiti per erogare mutui che consentirebbero agli enti locali una programmazione decente degli interventi e un respiro più largo rispetto ai debiti contratti. Ma in questo provvedimento le questioni erano altre. Intanto una sorta di deresponsabilizzazione totale. L'introduzione di una aggravante di pena connessa ad una sorta di si potrebbe definire quella che verrà introdotta oggi. Attraverso la delimitazione territoriale dei confini entro cui un reato, nel nostro Paese, si paga di più si cela un'idea del Paese e dei cittadini italiani ignobile. Siamo oltre la Costituzione. Siamo oltre il principio che davanti alla legge tutti sono uguali. Da oggi, se verrà convertito questo decreto-legge, alcuni cittadini italiani rischiano di essere trattati diversamente solo perché nati nel Sud d'Italia. E poi la questione degli interessi che ruotano intorno ai termovalorizzatori. Basterebbe fare due conti per verificare l'inutilità della concentrazione di alcuni di essi. Nel provvedimento non c'è nessun ragionamento o distinzione sulla gradazione dell'incentivazione, né rispetto alle Regioni, ne rispetto agli ATO, né considerando l'efficienza energetica di questi impianti, così come ci raccomanda l'Europa. Ancora una volta piccoli interessi industriali andranno a limitare lo sviluppo dell'energia rinnovabile, sottraendo risorse destinate alla ricerca, all'innovazione e all'uso di fonti pulite d'energia. Si può affrontare questo argomento - mi rivolgo alla maggioranza e al Governo - laicamente in Parlamento? Se per i termovalorizzatori c'è necessità di incentivi pubblici, si può decidere in maniera trasparente? E per fortuna si è riconosciuta la parte di biodegradabile all'interno del rifiuto indifferenziato. Ma il problema è più profondo: è politico e culturale. Si scontrano due visioni della questione ambientale, due modelli di società. Alcuni di noi ritengono che non disponiamo del diritto di utilizzare delle risorse ambientali a nostro piacimento. Alcuni di noi pensano che esista un diritto del futuro, futuro, dell'umanità che ancora non c'è, a vivere in un mondo meno contaminato, meno sfruttato, maggiormente sicuro. Alcuni di noi addirittura pensano che il Creato non ci appartenga. Ci sarà un motivo se anche sull'argomento specifico insistiamo sulla differenziata, sul riuso, sul riutilizzo, sul rinnovabile. La nostra non è una posizione ideologica, ma ideale sì. Non ci appartiene il mondo «usa e getta» al quale la posizione, quella sì ideologica, di alcuni di voi vorrebbe piegarci. Non ci appartiene una visione che non si vuole fare carico del destino dei nostri figli e di chi verrà dopo di noi. Incenerire, bruciare, distruggere per consumare e poi consumare e consumare. Con questa posizione non c'è futuro. E senza obiettivi eticamente motivanti, oserei dire dotati di senso religioso, diventa sempre più difficile governare un presente che sfugge di mano. Infine, questo è un decreto che dovrebbe servire a gestire una cronica emergenza. Sono d'accordo con quanti sostengono che è giunto il momento di sistematizzare la cronicità: vale anche per altri tipi di emergenza. Stabilisca il Parlamento una griglia di operazioni da compiere e di atti da produrre in presenza di emergenze. Altrimenti, sarà sempre un rincorrere, ogni volta e comunque, segmenti e particolarità che l'imprevisto comporta e dentro queste particolarità ognuno ci infila un pezzo di interessi che nulla hanno a che fare con l'emergenza, così come questa volta il decreto in esame non c'entra niente con i rifiuti di Napoli.

onorevoli colleghi e colleghe, anch'io ridurrò a pochissimi minuti, meno di quelli che sarebbero a mia disposizione, le mie considerazioni, chiedendo alla Presidente di lasciare agli atti il mio intervento. ARMATO *(PD)*. Il problema della raccolta e della gestione dei rifiuti dovrebbe essere - e purtroppo siamo ancora al «dovrebbe» - una grande questione di civiltà, una questione centrale in ogni programma di Governo moderno.

una parte dei cittadini del nostro Paese, tra l'altro quella parte già duramente provata dall'emergenza, ossia i cittadini della Campania. Campania. Non si è messo mano a un programma complessivo, generale e definitivo di gestione dei rifiuti e di risanamento ambientale, sia per la Campania che per il resto d'Italia; è stato già sottolineato come questo sia un problema che si sta ora aggravando

previsione di sanzioni a carico degli enti locali e dei Comuni in maniera decisamente più adeguata alla nostra Costituzione e soprattutto alla necessità di sostenere i Comuni nella battaglia per la differenziata e per un ambiente migliore. Ancorché migliorato, questo è comunque un decreto che su alcuni punti su alcuni punti è ancora troppo negativo; quei punti sono stati illustrati, si è detto della loro incostituzionalità.

che sarebbero dovute servire a recuperare il territorio, spesso martoriato nei decenni passati - e ben prima dei quattordici anni di commissariamento - dall'essere considerato lo sversatorio dei rifiuti, anche tossici, provenienti da tutta Italia.

I Governi successivi hanno solo attuato quello che si è messo in campo: i termovalorizzatori, l'individuazione dei CDR. Ricordo che quando fu individuato tra i CDR anche la mia area di residenza

quei milioni di ecoballe che, come ricordava il relatore, non potranno essere portate agli inceneritori, perché non sono secche, ma sono umide. Anzi, ora veramente non lo sono più, perché sono là da così tanti anni che sono piene di biogas.

Signora Presidente, colleghi senatori, in seguito all'invito alla brevità, svolgerò un intervento di pochi minuti, chiedendo alla Presidenza di lasciare agli atti il mio testo scritto.

chi commette un reato di tipo ambientale debba essere punito in maniera diversa, a seconda che lo commetta in Lombardia o in Campania. Inoltre, si è sottovalutata, circoscrivendo le sanzioni alle sole Regioni commissariate, la presenza della criminalità organizzata: le Regioni in emergenza sono quelle che hanno una presenza della malavita molto forte che non ha difficoltà ad esercitare quelle inadempienze nelle Regioni limitrofe e cioè in zone franche, in un limbo dove tutto è meno grave. Un'altra parte del disegno di legge di cui non condividiamo assolutamente niente è l'articolo 9, in cui si introduce un'incentivazione per la costruzione di impianti di incenerimento ancora una volta in maniera surrettizia. Di fatto, non viene operata una distinzione nell'incentivazione, né rispetto alle Regioni, né considerando l'efficienza energetica di questi impianti, così come raccomandato nell'ultima direttiva quadro europea sui rifiuti. Approfittando di questo disegno di legge, il Governo ha deciso di estendere le tariffe agevolate CIP6 ai termovalorizzatori, nei quali viene bruciata anche la componente inorganica dei rifiuti (che dovrebbe in teoria essere differenziata e riciclata) insieme ai rifiuti organici, che sono quelli realmente rinnovabili. Oltre a rappresentare un assurdo per la conduzione delle politiche ambientali, le mosse del Governo produrranno un aggravio dei costi A nessuno, infatti, deve sfuggire che gli incentivi per le fonti rinnovabili sono finanziati dalle bollette dell'energia elettrica e l'assimilazione dei termovalorizzatori alla categoria degli degli impianti rinnovabili produrrà un significativo aumento dei costi per tutti i cittadini italiani. Forti dubbi, tra l'altro, sussistono per quanto riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria. Vorrei ricordare un dato relativo alle circa 160 procedure di infrazione pendenti per l'Italia, di cui ben 43 - cioè un quarto - sono relative all'ambiente Di queste, ben 12 sono determinate dal mancato rispetto del nostro Paese della normativa europea in materia di rifiuti. Un inciso, essendo io senatrice farlo anche sulla mia Regione. In Calabria dal lontano 1997 la partita ambientale è affidata alla gestione di un commissario delegato. undici anni di gestione commissariale i problemi anziché essere risolti si sono acuiti: non è stata praticata un'attività di programmazione per individuare strategie e strumenti per dare una giusta ed equilibrata risposta a tutte le aree territoriali. L'esempio più eclatante dello squilibro è Crotone, divenuta la pattumiera della Calabria e per anni anche di Napoli. A Crotone, dove ancora confluiscono i rifiuti di 27 comuni della provincia di Cosenza, la gestione dello smaltimento è nelle mani di privati a cui è stato negato tra l'altro il certificato antimafia per problemi di tipo mafioso. Sempre a Crotone, il commissario delegato per l'emergenza ambientale, il 3 luglio 2001, ha approvato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con alimentazione a rifiuti non pericolosi e pericolosi; un impianto di termovalorizzazione che ha la capacità di trattare 22.000 tonnellate all'anno di rifiuti speciali; in aggiunta, vi è un impianto di inertizzazione che può trattare 12.000 tonnellate all'anno di rifiuti liquidi, solidi pastosi, fanghi e melme dell'industria petrolifera e petrolchimica. Lo scorso anno il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria ha concesso una proroga per il completamento del progetto del termovalorizzatore a Crotone. L'impianto è stato quasi ultimato e presto entrerà in funzione, nonostante non abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Data la persistente situazione di emergenza, non è escluso che presso il termovalorizzatore di Crotone possano confluire rifiuti provenienti dal resto della Regione e da altri territori nazionali. situazione di gravità che esiste in questa città per la mancata bonifica dell'ex sito Pertusola, si capisce come alcuni territori siano particolarmente in difficoltà per quanto riguarda la salubrità ambientale e la salute dei cittadini.

alle regole, soprattutto in materia ambientale, perché affrontare un'emergenza oggi potrebbe produrre danni per l'ambiente e la salute dei cittadini domani. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, intervengo innanzitutto perché ritengo opportuno e oltremodo doveroso, da cittadino della Campania ancorché senatore della Repubblica, rendere atto al Governo del presidente Berlusconi per l'impegno straordinario assunto e sostenuto con costante determinazione e coraggio a favore di una Regione che ha rischiato la catastrofe. Ben conoscendo la storia del nostro Paese e le diverse tragedie che ne hanno segnato il cammino, non possono non sovvenirmi alla mente le metodologie, le logiche e i tempi con i quali e nei quali sono state affrontate, nei decenni passati, le gravi relative emergenze; penso al terremoto del Belice, del Friuli e della mia Irpinia. Grande e diffusa solidarietà, enorme impegno di tutti, istituzioni e cittadini, ma su tutto troppo spesso tanta confusione e tanto tempo sprecato; anni e anni, decenni trascorsi a realizzare programmi di ricostruzione paradossalmente ancora oggi in corso, e tanto denaro al vento. La Campania, vorrei ricordarlo (ma credo che le immagini che appena qualche mese fa hanno girato il mondo siano impresse indelebilmente nella nostra mente e lo saranno per sempre), era arrivata all'orlo del precipizio. L'emergenza rifiuti, che poi era ed è l'emergenza ambientale, ha rischiato di trasformarsi - e non credo di esagerare - in disastro sanitario. Un'emergenza, aggiungerei, che ha rischiato di innescare un irreversibile stato di sollevazione popolare ed insorgenza. Penso al caso Pianura o alla protesta di Chiaiano: quartieri nei quali la portata dei disordini e il tentativo del malaffare di infiltrarsi *pro domo sua* nei gangli della protesta ha rischiato di trasformare il malcontento in sollevazione popolare. Se oggi possiamo dire di averla scampata bella, lo dobbiamo alla volontà, alla prontezza e all'efficienza di un Governo e di un *Premier* che, senza perdersi in ideologismi di sorta, ha compreso la gravità della situazione affrontandola di petto ben intuendo le difficoltà cui andiamo incontro, ben conoscendo il livello di resistenza, non solo delle popolazioni ma anche di certa irresponsabile politica locale. Oggi appare lontana l'eco di quelle immagini e l'acuzie di quell'emergenza è acqua passata. La capacità e il quotidiano impegno del sottosegretario all'emergenza rifiuti, dottor Bertolaso, hanno consentito alla Campania il rientro di un'emergenza le cui conseguenze hanno attraversato l'intero Paese. I risultati conseguiti a tutt'oggi, va sottolineato, sono lusinghieri, anche considerati i tempi. L'impegno assunto, cioè l'uscita della Campania dalla fase acuta dell'emergenza, è stato mantenuto e la strada che conduce alla normalità, alla fine del commissariamento, ad una corretta gestione dell'intero ciclo rifiuti è stata intrapresa, seppur tra mille oggettive difficoltà. Ed è proprio in ossequio a queste considerazioni, nella necessità di realizzare una corretta logica di sistema impermeabile al malcostume, al malaffare, che incentivi la cultura del rifiuto come risorsa, colleghi del Senato, che va inquadrato l'atto che oggi è sui nostri banchi: misure specifiche per la soluzione definitiva, ultima, della crisi. E così, colleghi senatori, con queste norme si va e si andrà verso la soluzione definitiva della crisi. Una crisi, aggiungerei, che se da un lato sembra finalmente voler abbandonare la Campania, dall'altro sembrerebbe voler esplodere purtroppo in altre Regioni. In questo senso, se in Campania, dopo oltre 14 anni si è riusciti a cambiare registro è perché le misure messe in campo in questi pochi mesi, per l'efficacia che hanno saputo dimostrare, per la qualità degli uomini che le hanno volute ed attuate, sono considerate un modello di riferimento e, per quanto perfettibile, un esempio da seguire laddove, purtroppo, si rendesse necessario. Misure specifiche, dicevo, per la soluzione definitiva. Misure che, esplicati gli effetti e stabilizzati gli obiettivi, potranno finalmente scrivere con inchiostro indelebile la parola fine al commissariamento, ribadisco, dopo oltre 14 anni. Misure che hanno il merito, in una attenta e coerente condizione di *work in progress* rispetto alle norme straordinarie già messe in campo nei mesi scorsi, di individuare quelle ulteriori o sopraggiunte criticità che in qualche modo costituiscono un freno al processo di normalizzazione del ciclo dei rifiuti. Norme necessarie, rilevo, che tengono conto di esigenze imprescindibili e che hanno il pregio di un più diretto coinvolgimento del cittadino che questa volta è parte utile ed incentivata di uno dei tasselli principali dell'intero ciclo rifiuti: la raccolta e il trasporto di singole tipologie di imballaggio, come il vetro o l'alluminio, presso le aree attrezzate e autorizzate. Norme che premiano chi si fa parte diligente, attiva e responsabile e che, di contro, intervengono con sanzioni penali speciali con chi deposita o smaltisce abusivamente rifiuti ingombranti o tossici. Norme, per portare qualche esempio, che non fanno sconti alle amministrazioni locali inefficienti o, peggio, inerti. Norme, ancora, che fanno dell'educazione ambientale materia di studio nelle scuole. Ma, soprattutto, norme che estendono gli importanti incentivi del CIP6 alla realizzazione dei termovalorizzatori riconoscendoli quali impianti assimilati alle fonti energetiche rinnovabili. insomma, che dovrebbero tagliare definitivamente la testa al toro finanche accelerando quel percorso virtuoso che dovrà consentire alla Campania, per la prima volta nella sua storia, di attrezzarsi utilmente ed efficacemente per una gestione razionale e di prospettiva dei suoi rifiuti. Ma è a questo punto, signora Presidente e colleghi, e cioè nel delicato passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria, di competenza regionale, che sarà necessario scongiurare il rischio che si abbassi il livello di guardia. All'attuale normativa campana sul ciclo dei rifiuti, che ritengo fortemente ideologizzata, fortemente politica e scarsamente efficace, riconosco comunque il merito di aver individuato un principio di fondo: l'autonomia su base provinciale dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un principio teso a scongiurare la malaugurata condizione di Province che, pur producendo un monte rifiuti modesto, si vedono accollare sui propri siti, sui propri impianti ciò che altre Province, per incapacità e inefficienza, per negligenza o, peggio, premeditatamente,

infrastrutturali esistenti tra una Provincia campana e l'altra, ma che ha comunque prodotto uno sbilancio di trattamento tra Province virtuose e Province tutt'altro che virtuose. Comprendiamo tuttavia le necessità e le inevitabilità che possono sorgere nei casi di emergenza acuta, ma auspico, da cittadino di una tra le Province in questo senso più virtuose e purtroppo maggiormente sacrificate, almeno nella fase conclusiva del percorso che dovrà portare al passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria, e che, allorquando si riterranno maturi i tempi per la gestione ordinaria, tale principio possa valere con il massimo del rigore. Al Governo chiedo di fare il possibile affinché il principio dell'autonomia su base provinciale dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti possa trovare già oggi condizioni favorevoli. Così come auspico, e mi avvio alla conclusione, che allorquando - spero il più presto possibile - sarà superata la fase commissariale, il Governo, pur nei limiti delle sue competenze, vigili con la massima attenzione

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parete di nulla osta sul testo, nel presupposto che all'articolo 8 non sia superato il limite di 35 unità dì personale e che i contributi compensativi per gli enti locali, di cui all'articolo 9-*ter*, siano individuati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2-*ter*.0.1, 6.22, 8.1, 9-*ter*.2, 4.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Con la premessa che l'argomento andrebbe trattato con la Commissione attività produttive, viste le

G102, con la permessa che in questo caso l'ordine del giorno andrebbe a creare una situazione di sovrapposizione alle attività già svolte dalle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria, mi rimetto al Governo. Anche nel

lo accoglierei come raccomandazione.

l'emendamento 4.200 si illustra da sé. Esso risponde a ragioni di diritto, ma anche di buon senso, per evitare che i contratti in corso al momento della costituzione della società

*(PD)*. Signora Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione, quella del rappresentante del Governo e naturalmente quella dei colleghi senatori sull'emendamento 5.2, che per il Partito Democratico si è reso necessario verosimilmente soltanto per consentire al Governo di esplicitare meglio la propria volontà. Vorrei in particolar modo, se ciò non dovesse significare una forma di involontaria trascuratezza nei confronti degli altri colleghi, rivolgere una preghiera di attenzione ai colleghi della Commissione difesa dei quali, signora Presidente, conosco bene, peraltro alla pari degli altri, la sensibilità.

armate. Le Forze armate, secondo la lettera del decreto, dovrebbero essere impiegate per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Mi verrebbe da chiedere, e comunque glielo chiedo, se, quando si parla di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, si vuol dire che le Forze armate sono chiamate a svolgere attività di sorveglianza su dove e come i cittadini si liberano dei rifiuti; se sono chiamate ad occuparsi della raccolta dei rifiuti;

decreto, ma di essere chiari e di specificare se, quando si parla di controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, per caso non si intenda trasformare *tout le Forze armate in operatori ecologici, sia che raccolgano materialmente le buste di nettezza urbana sia che guidino quei mezzi.

Non credo che sotto Natale questo Governo, anziché la divisa tradizionale che con grande dignità le Forze armate indossano, voglia regalare loro una divisa di operatore ecologico. chiedo al Governo di sapere se, in luogo di un eventuale parere contrario a questo emendamento, ci fosse la disponibilità ad accoglierlo come ordine del giorno.

Trattandosi infatti di un diritto temporaneo, collegato ad una norma costruita sulla base di un atto amministrativo che ne regge i presupposti, e che potrebbe essere tra l'altro collegato ad un atto regolamentare, ad un'ordinanza, piuttosto che ad un

Insisto ancora una volta perché almeno la normativa, per una ragione di omogeneità, sia estesa a tutto il territorio nazionale.